L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

il 20 novembre 1989 venne approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; che è giustamente considerata la pietra miliare per la tutela delle bambine e dei bambini di tutto il mondo, in quanto riconosciuti quali soggetti di diritti a pieno titolo. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che mi onoro di presiedere, si è di fatto costituita proprio la settimana scorsa, quindi per noi non c'è occasione migliore di questa ricorrenza per iniziare il nostro mandato. Ogni anno, in ricordo di quel momento storico, celebriamo, proprio il 20 novembre, la Giornata internazionale del fanciullo, una data simbolica, che richiama tutti noi cittadini, ma soprattutto il legislatore, a fare i conti con quanto è stato fatto in sostegno e in difesa dei bambini e soprattutto con quanto ancora si debba fare sul fronte dei diritti dei bambini e degli adolescenti, primo su tutti il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; ma anche il diritto di espressione, di partecipazione, di considerazione e soprattutto di ascolto. Ciò su cui desidero richiamare la vostra attenzione è, in particolare, un principio sancito dalla Convenzione, che ormai troppo spesso è ignorato, se non consapevolmente negato: quello del superiore interesse del bambino. Sottolineo in quest'Aula l'importanza di questo principio, che dovrebbe essere la bussola per orientare gli interventi del legislatore non solo in materia di diritto di famiglia, ma ogni qualvolta si assumono le decisioni che andranno a incidere direttamente sulla vita dei nostri figli o dei nostri nipoti. Cosa è bene per i nostri bambini? Siamo certi di rispondere a una loro esigenza, di contribuire alla loro crescita, di fare, in altri termini, il loro interesse? Molto è stato fatto da parte del Parlamento. Penso, ad esempio, alla recente approvazione della legge sul cyberbullismo, ma purtroppo non è stato sempre così. Vedete, colleghi, abbiamo una grandissima responsabilità: attraverso i nostri interventi contribuiamo a formare le donne e gli uomini di domani a costruire il loro futuro. Cito velocemente solo alcuni dati, purtroppo impietosi, che ci confermano che l'Italia non è un Paese per giovani. Secondo l'ISTAT, nel 2017 i nati sono stati più di 450.000; oltre il 12 per cento dei bambini e adolescenti italiani vive in condizioni di povertà assoluta;

Dati che vanno necessariamente accostati, che fotografano una realtà amara, che vede tanti minori vincolati alle condizioni di disagio delle loro famiglie, impossibilitati a emanciparsi da esse, costretti ad abbandonare la scuola e a vedere negato il proprio diritto a essere bambini.

Il mio auspicio è che in questa legislatura ci sia un approccio responsabile da parte di tutti i partiti, in modo totalmente trasversale,

che la nostra voce vada soprattutto a proteggere quei bambini che voce non hanno e con maggiori difficoltà.

I bambini non riconoscono il colore della pelle, non vedono le differenze di censo, non vedono nessuna differenza né discriminazione; imparano le differenze soltanto tramite gli adulti. Ecco io credo che avremmo molto da imparare dai bambini in questo e probabilmente dovremmo riuscire anche noi, quando ci occupiamo di bambini, ma anche quando ci occupiamo di altro, a guardare il mondo proprio «con gli occhi trasparenti di un bambino», come diceva una bellissima canzone. Grazie a tutti. *(Applausi dai

passiamo direttamente al successivo punto all'ordine del giorno, che reca discussione di ratifiche di accordi internazionali.

il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2017 tra il nostro Paese e il Giappone sul trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa. Il testo riproduce i contenuti dell'Atto Senato 2971, esaminato dalla Commissione affari esteri del Senato nel dicembre 2017, provvedimento che non poté tuttavia completare il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura. L'Accordo in esame si compone di un preambolo e di sette articoli ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui consolidare la collaborazione in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi, per agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e produzione congiunta, anche a beneficio delle industrie nazionali di difesa, nel quadro del comune impegno per contribuire alla pace e alla stabilità internazionale. Il testo in esame, dopo aver enunciato gli scopi dell'intesa, istituisce un Comitato congiunto preposto a definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti e dispone l'obbligo per le parti di utilizzo delle dotazioni scambiate nel rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, vietandone altresì il trasferimento a terzi senza previo consenso della parte che ha originato il trasferimento stesso. I successivi articoli disciplinano il trattamento di informazioni e documenti classificati, precisano che le misure dell'Accordo e di quelle da esso derivanti saranno attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna parte, definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative ed enunciano le disposizioni relative all'entrata in vigore, all'eventuale modifica e alla denuncia del testo. Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di cinque articoli, che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore. Con riferimento infine agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 4.529 euro ad anni alterni a decorrere dal 2018, imputabili alle sole spese di missione dei rappresentanti della Difesa per la loro partecipazione alle riunioni del Comitato congiunto in Giappone. La Commissione bilancio, nel formulare sul provvedimento in esame un parere non ostativo, lo ha fondato sul presupposto che a eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi. Evidenzio, infine, come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Con queste premesse propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dall'Assemblea.

Mi perdonerete se non sospendo la seduta per due minuti ma li lascio trascorrere, in modo da dare a tutti la possibilità di un esame di coscienza, di riflettere. Due minuti fanno sempre bene. Ecco, ora possiamo procedere.

del ministro *pro tempore* Pinotti a Tokyo, in un'importante missione che ha sancito un salto di qualità nelle relazioni, dal punto di vista della difesa, tra il Giappone e l'Italia. Voglio mettere in evidenza due aspetti importanti: questo è un Accordo che è stato fatto nell'ambito della collaborazione con la NATO, quindi nel pieno rispetto dei nostri accordi internazionali e della Carta delle Nazioni Unite, e non solo ha a che fare con lo scambio di informazioni e di collaborazione fra i sistemi di difesa del Giappone e del nostro Paese, ma inserisce uno schema di riferimento per la collaborazione in ambito industriale per

Da questo punto di vista, lo salutiamo con favore. La ratifica non ha niente a che fare con la promozione di una maggiore vendita di armi all'estero; sappiamo che ci sono normative molto rigorose da questo punto di vista. È un tema che abbiamo affrontato anche all'interno della Commissione, dove c'era stato un fraintendimento, in particolare con il Gruppo del MoVimento 5 Stelle che chiedeva di rallentare rispetto alla ratifica, ma poi fortunatamente si è risolto e abbiamo potuto procedere.

ma questo sistema di alleanze oggi incontra alcune criticità rispetto al passato, soprattutto tra Giappone e Cina nel Mar Cinese meridionale e occidentale, laddove ci sono isole contese tra i due Stati. C'è poi l'atteggiamento degli Stati Uniti, che è cambiato rispetto alle amministrazioni precedenti, sia di Bush che di Obama; vi sono la nuova politica protezionistica, i dazi e l'apertura nei confronti della Nord Corea. Nonostante quindi sia sempre stato alleato degli Stati Uniti (il rapporto fra Shinzo Abe i *leader* precedenti è sempre stato molto forte), con la nuova politica statunitense il Giappone ha bisogno di sentirsi rassicurato e di costruire alleanze più larghe con l'Europa, con la NATO più in generale e, dentro la collaborazione con i Paesi europei, una relazione speciale con il nostro Paese. Questo apre spazi di collaborazione importante per la nostra

a questo trattato e speriamo che sia un'occasione in più di collaborazione positiva con un Paese come il Giappone, con cui abbiamo già ottime relazioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare ratifica un Accordo lungamente atteso dalle parti, Accordo di rilevanza strategica per l'industria italiana, riguardante il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia avanzata nel settore della difesa. Tale Accordo si inserisce all'interno di un percorso di collaborazione iniziato nel 2012, con la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti tra i rispettivi Ministri della difesa, che stabiliva la comune intenzione di avviare un dialogo bilaterale in campo militare e che ha condotto alla stesura, di un *memorandum* di intesa tra i due Ministeri in merito alla cooperazione e agli scambi nel settore di propria competenza, al fine di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza. Nello specifico, l'Accordo si compone di sette articoli, preceduti da un breve preambolo che richiama l'entrata in vigore, nel 2016, di un altro Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone e riguardante la sicurezza delle informazioni, nonché il Programma di cooperazione stipulato tra il Giappone e la NATO nel 2014. In particolare, i due Paesi intendono agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e produzione congiunta, anche a beneficio delle proprie industrie operanti nel settore della difesa. L'Accordo è stato concluso nel pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione: il nostro Paese, infatti, si colloca nel quadro del comune impegno per contribuire alla pace ed alla stabilità internazionale e nel rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. La cooperazione mira a valorizzare i rapporti a livello tecnico-industriale con un Paese, il Giappone, terza potenza economica del pianeta, con cui vantiamo solidi legami culturali e di grande rilevanza economica e tecnologica. Nell'ottica di questa collaborazione, e nel rispetto rigoroso di quanto disposto dal nostro ordinamento, incluse le norme e le procedure in materia di esportazione di materiali di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990 e dell'articolo 537-*ter* del codice dell'ordinamento militare e del regolamento di cui al decreto del verrà consentito al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrative finalizzate a favorire, da parte del Governo giapponese, l'acquisizione di materiali per la difesa prodotti dalla nostra industria nazionale. La sottoscrizione dell'Accordo faciliterà, inoltre, la costituzione di partenariati nel settore, anche in direzione dei mercati di Paesi terzi. L'Accordo con un Paese situato in un'area del Pacifico soggetta a profonde trasformazioni geopolitiche riveste una particolare importanza per gli interessi dell'Italia. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

l'Accordo con il Governo giapponese è particolarmente importante, perché ha lo scopo di gettare le basi per una cooperazione italo-nipponica nello scambio di equipaggiamenti e tecnologia di difesa. Come illustrato dal collega precedentemente, il testo dell'Accordo, infatti, non determina specificatamente dei trasferimenti, ma funge da quadro per gli interscambi futuri, che verranno concordati fra le parti. Inoltre, la sua attuazione consentirà di sostenere le industrie nazionali di difesa, facilitando la creazione di partenariati industriali anche in direzione dei Paesi terzi. Questo è un punto molto importante. Infatti, è inutile nascondersi che solo attraverso la cooperazione con Paesi pacifici come il Giappone è possibile aumentare la nostra facoltà di scegliere gli interlocutori in un settore complesso come quello dei trasferimenti di armamenti e, in alcuni casi, sapere dire anche di no a qualche Stato o a qualche organizzazione che eventualmente ritenessimo poco affidabile. In questo Accordo due sono gli elementi più importanti: il primo, la creazione di un Comitato congiunto al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa da trasferire, che permette al nostro Ministero della difesa di adeguare meglio i progetti in corso, la cui composizione, come sapete, è garante degli interessi dei rispettivi Ministeri della difesa. Il secondo punto importante, l'articolo 3 - permettetemi di dire - ha una rilevanza particolare, in quanto fa esplicito riferimento al rispetto del diritto internazionale, vincolando le parti ad utilizzare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa, eventualmente scambiati rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite e gli ulteriori scopi specificati nell'intesa autorizzante il trasferimento. Inoltre, vieta il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza il previo consenso della parte mittente, in ottemperanza della nostra legge n. 185 del 1990, che, nonostante non sempre abbia impedito vendite quantomeno immorali, rappresenta comunque un punto di riferimento a livello internazionale. Il Giappone, come tutti sappiamo, è un Paese pacifico, e la cooperazione in questo caso ha il solo scopo di potenziare e migliorare la difesa del Paese da eventuali minacce, non certo di essere impiegata in qualche guerra umanitaria, come si dice oggi. Per questo non abbiamo da temere, sulla base delle informazioni in nostro possesso, anche a partire dalla storia recente del Paese e dall'equilibrio delle forze in campo, che queste tecnologie e gli effetti che ne deriveranno possano essere utilizzati per nuocere ad altri Paesi o per violare i diritti umani. conclusione, credo che questo sia un Accordo davvero vantaggioso per entrambe le parti. Infatti, sia l'Italia che il Giappone rappresentano due punti di riferimento nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, in campo civile e militare. Per le ragioni sopra citate e per l'interesse strategico della nostra difesa e del nostro Paese, dichiaro all'Assemblea il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle sulla ratifica dell'Accordo per il trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa con il Giappone. *(Applausi

dire che condivido il fatto che abbiamo una *partnership* speciale con il Giappone, e mi compiaccio con il Governo di aver portato - mi rivolgo al sottosegretario Picchi - il provvedimento all'attenzione del Senato per l'approvazione. È positivo perché non potevamo più far aspettare il Giappone. Questo Accordo fa parte di un tassello di relazioni che abbiamo con questo Paese, che - non dimentichiamocelo - pur essendo tanto distante da noi, è un Paese con cui

Come si evince dalla relazione introduttiva, il testo al nostro esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente al solo Accordo con il Montenegro, il disegno di legge di ratifica di numerosi accordi internazionali bilaterali proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (Atto Senato 2813) che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, senza peraltro poter completare il proprio *iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura. Ricordo che il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo, è divenuto indipendente nel 2006, e da allora, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che potrebbero derivarne, si è avviato con decisione sulla via dell'integrazione europea ed atlantica. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione di fatto dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012. Ad oggi, su un totale di 35 capitoli negoziali, ne risultano aperti 31, tre dei quali già provvisoriamente conclusi. Il Montenegro considera peraltro l'Italia come un punto di riferimento essenziale per il suo percorso di avvicinamento all'Unione europea, anche in ragione dei forti legami culturali esistenti tra i due Paesi. La cooperazione nel settore culturale e dell'istruzione ricopre quindi un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Lo scopo principale dell'Accordo in esame è in effetti propriamente quello di consolidare e di armonizzare i legami culturali esistenti e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro. Il provvedimento, in particolare, che si compone di un preambolo e di diciotto articoli, oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di borse di studio faciliterà la cooperazione anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e demo-etno-antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. che prevede anche una stretta collaborazione nei campi dell'archivistica e biblioteconomia, dell'informazione, dell'editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili, rappresenterà altresì un valido strumento anche per la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali. Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, agli impegni finanziari, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore. oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati complessivamente in 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.

in esso contenuto rappresenta la conclusione di un percorso, intrapreso nella scorsa legislatura, e di un cammino unito tra l'Italia e il Montenegro. Il relatore ha detto alcune cose importanti relativamente ai rapporti tra Italia e Montenegro, un Paese che in questi anni sta compiendo un percorso molto importante e quasi d'esempio perché, dopo esser stato protagonista di una indipendenza dalla Serbia senza sparare neanche un colpo (quindi un esempio quasi unico nei Balcani nella storia degli ultimi secoli), ha poi intrapreso con grande decisione la strada dell'integrazione in Europa sotto vari profili,

dal percorso d'integrazione nell'Unione europea. Il senso di questo desiderio di entrare in Europa è stato dato immediatamente perché, appena divenuto indipendente, il Montenegro ha adottato l'euro. l'euro. Questo è stato quindi un segnale forte di voler andare nella direzione dell'integrazione europea. Spesso si parla di allargamento dell'Unione, ma va considerato un aspetto. Noi vogliamo allargare l'Unione non a Paesi euroscettici,

balcanici la scelta del Montenegro non è stata facile, ma contrastata e ha anche avuto delle ripercussioni interne, soprattutto nei rapporti con altri Paesi limitrofi.

sul proprio territorio decine di migliaia di profughi di quel Paese e tutto questo lo ha fatto con un grande senso di solidarietà e disponibilità. La terza cosa che voglio, infine, sottolineare è legata agli interessi dell'Italia nei confronti della penisola balcanica. Se esiste una propensione dell'Italia ad avere un'influenza economica su una importante regione dell'Europa,

decadrà a tutti gli effetti l'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale socialista di Jugoslavia che venne firmato a Roma il 3 dicembre del 1960. rappresenta la base giuridica necessaria ad avviare iniziative e progetti di scambio culturale tra i nostri Paesi e dà esecuzione all'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione sottoscritto dall'Italia e dal Montenegro grazie. che l'Italia, però, ha forti ragioni e legami culturali con questo Paese ed è un punto di riferimento essenziale per il percorso di avvicinamento all'Unione europea del Montenegro. Lo scopo principale di questo Accordo, nel rispetto della normativa nazionale, dell'ordinamento europeo e degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è in effetti propriamente quello di consolidare e di incrementare tali legami. Si è parlato poc'anzi di provvedimenti che promuovono iniziative a livello universitario e scolastico, dell'offerta di borse di studio, della diffusione nelle scuole e nelle università montenegrine della lingua e della cultura italiana: si tratta di aspetti estremamente importanti. In conclusione, questo Accordo prevede una stretta collaborazione anche nei campi dell'archivistica, dell'informazione e dell'editoria, rappresentando altresì un valido strumento anche per la protezione dei diritti d'autore, tanto attesi dai nostri imprenditori. Per queste ragioni,

Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, da più di duemila anni l'Italia e il Montenegro sono indissolubilmente legati da comuni radici culturali. Già l'impero romano, per circa cinquecento anni, aveva annesso il Montenegro all'Urbe. Mi dilungherei oltremodo se elencassi, in uno spazio temporale lunghissimo, il legame fra i due Paesi, ma per meglio fotografare la storia recente vado direttamente al secolo direttamente al secolo scorso, quando i rapporti si rinforzarono ulteriormente, con il matrimonio tra Vittorio Emanuele III, re d'Italia, e la principessa Elena di Montenegro. Questa millenaria amicizia non si interruppe nemmeno nel biennio 1918-1920, quando l'Italia, unico Paese europeo, si oppose alla cancellazione dell'indipendenza del Montenegro. La vicinanza culturale risultò addirittura più effervescente sotto il regime di Tito. Solo con la frantumazione della Jugoslavia i rapporti videro un appannamento, causato perlopiù dalla forte pressione delle cancellerie europee, che erroneamente puntarono ad un asse privilegiato con Belgrado. Per qualche anno la quasi totalità della comunità internazionale ha considerato il Montenegro, inclusi i governanti, come un Paese dedito al contrabbando di sigarette e rifugio di molti malavitosi italiani. Fu indagato per questo anche l'allora capo del Governo, Djukanovic infatti molte procure italiane lo iscrissero nel registro degli indagati. Il corso dell'attività investigativa dimostrò poi l'estraneità ai fatti, ma si acclarò che effettivamente le coste montenegrine furono usate come piattaforma operativa dai contrabbandieri balcanici e dai mafiosi italiani. Oggi quella rotta del tabacco risulta essere completamente smantellata, tuttavia qualche attento osservatore politico si è spinto a dire che le indagini a carico di Djukanovic furono solo formidabili accuse per screditare il neogoverno montenegrino, colpevole di essersi discostato troppo da Belgrado. In sostanza, millenni di amicizia e di scambi culturali furono bruciati in un decennio di cecità politica e direi anche di scarso realismo. Solo dal 3 giugno 2006 il Montenegro è diventato Stato indipendente, internazionalmente riconosciuto, e dal 2017 è il ventinovesimo membro della NATO, un Paese saldamente stabile, con un'economia in espansione, sia per quanto riguarda il turismo che le infrastrutture. Non può certo sfuggire che quel Paese oggi offre importanti possibilità di investimenti in infrastrutture stradali e per la rete ferroviaria. Anche la valorizzazione turistica potrebbe apparire conveniente per gli investitori italiani, considerando che il Paese risulta ancora poco conosciuto. Infatti, solo il 2 per cento dei turisti che visitano lo Stato adriatico proviene dall'Italia. Faccio riferimento a questi aspetti ben sapendo che l'Accordo oggetto di ratifica prevede la cooperazione culturale e di istruzione, ma proprio per questo non possono essere slegati con tutte le intese che, inevitabilmente, si andranno ad intrecciare. Per tutti questi aspetti la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, siglato a Roma il 15 aprile del 2014, saranno prodromiche rispetto a futuri e vantaggiosi rapporti. Pertanto, il MoVimento 5 Stelle non può che esprimere un voto favorevole.

tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Laos nel febbraio 2003. L'Accordo, composto da tredici articoli, si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione bilaterale, e di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, fornendo al contempo una risposta alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia che emerge nel Paese asiatico, ma offrendoci l'opportunità di allargare i nostri orizzonti economici e culturali anche in Asia, non solo quando si parla di delocalizzare imprese italiane. In particolare l'Accordo, dopo aver stabilito i princìpi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione, afferma la volontà delle due parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori e di mostre,

c'era brusio. Il testo prevede, altresì, che le attività di cooperazione scientifica e tecnologica si realizzino attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l'organizzazione di convegni, seminari e di altri eventi, nonché mediante la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di attività di addestramento e aggiornamento professionale. L'Accordo punta, inoltre, a promuovere la collaborazione nei campi archeologico e antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale, nonché la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e *post*-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche, oltre a prevedere l'impegno, nei limiti della disponibilità dei fondi, per l'erogazione di borse di studio per studenti e laureati per studi e ricerche a livello universitario, *post*-universitario o presso altre istituzioni accademiche nel campo delle belle arti, dell'archeologia e della linguistica. Il disegno di legge al nostro esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente al solo Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Laos, il testo di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, ma non vide completato il proprio *iter* di esame, nonostante la Commissione si fosse prodigata nell'approvazione di decine di accordi di cooperazione militare con Stati spesso in guerra o ai confini di grossi conflitti, tuttora in corso, e su cui credo sia necessario tornare per verificarne la compatibilità con la legge n. 185 del 1990. Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore. Signor Presidente, credo che il nostro Paese possa finalmente dare corso ad una nuova forma di relazione che superi i limiti del neo colonialismo, soprattutto con quei Paesi che hanno vissuto la tragedia del colonialismo e della guerra. Ricordo che il Laos è un Paese del Sud-Est asiatico di oltre 6 milioni di abitanti, privo di sbocco al mare e che si sviluppa lungo il corso del fiume Mekong, in un'area geografica della penisola indocinese stretta fra il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia, il Myanmar e la Cina. Protettorato francese dal 1893, indipendente dal 1954, il Laos ha subìto pesantemente l'aggressione degli Stati Uniti in Vietnam: sul Laos tra il 1964 al 1973 vennero sganciati due milioni di tonnellate di ordigni esplosivi e ancora oggi ci sono circa 80 milioni di bombe da disinnescare che continuano a mietere vittime tra persone e animali. Si pensi che ancora oggi, ogni anno più di 300 persone restano vittime di queste esplosioni, la metà muoiono e di questi la maggioranza sono bambini.

fino al 1997, anno in cui ha optato per l'adesione all'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), avviandosi sulla strada della piena integrazione regionale e internazionale. Dal 2013 è entrato ufficialmente a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Il Paese ha un'economia prevalentemente rurale e vanta una grande disponibilità di corsi d'acqua, condizioni che potrebbero favorire la cooperazione agricola con l'Italia e dare ulteriori sbocchi economici per le nostre imprese agricole, che vivono una fortissima crisi economica. Altri settori su cui potrebbero nascere proficue collaborazioni sono quelli idroelettrico e minerario, veri volani dell'economia nazionale, anche grazie agli investimenti diretti esteri provenienti in particolare dalla Cina e dall'Australia.

sono convinto che i frutti di questo Accordo saranno reciproci. Inutile nascondersi che l'Italia vive una forte crisi di isolazionismo internazionale, che privilegia i nostri *partner* storici, ma ignora del tutto le nuove opportunità che il multilateralismo ha creato, soprattutto in Asia. Per questi motivi chiedo ai colleghi di supportare questo Accordo votando a favore.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Laos è un Paese del Sud-Est asiatico con oltre 6 milioni di abitanti, privo di sbocco sul mare e che si sviluppa lungo il corso del fiume Mekong, in un'area geografica della penisola indocinese stretta fra il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia, il Myanmar e la Cina. Il Laos è stato un protettorato francese dal 1893 ed è diventato indipendente nel 1954. Nel dicembre 1975 è diventato una Repubblica democratica popolare e dal 1997 aderisce all'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, avviandosi sulla strada della piena integrazione regionale e internazionale. Dal 2013 il Laos è entrato ufficialmente a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, con un'economia prevalentemente rurale che vanta una grande disponibilità di corsi d'acqua, - queste - che potrebbero favorire anche la cooperazione agricola con l'Italia e dare ulteriori sbocchi economici alle nostre imprese agricole. Con il disegno di legge che ci accingiamo a votare si avvia il processo di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra l'Italia e il Laos. Questa ratifica si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione tra i due Paesi ed è per questo che il Partito Democratico è favorevole. Dare priorità alla politica di accordi di cooperazione internazionale volti a facilitare l'interscambio economico e culturale, la tutela dell'ambiente e lo scambio di tecnologia è un fatto molto positivo. Credo che sia una direzione giusta per poter portare sviluppo all'Italia, ma da sola non basta. Infatti, bisogna lavorare - anche e soprattutto - su una politica estera e di sviluppo economico che miri molto di più all'internazionalizzazione dell'Italia nel mondo. Gli accordi sono il primo passo. Per un Paese che vuole definirsi civile e guardare con spirito positivo al futuro, la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, a tutti i livelli, è un'opportunità per rivolgersi al mondo e aprire i propri confini. Come sottolinea il testo che ci accingiamo ad approvare, si cerca anche di fornire una risposta alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia in Laos: una richiesta di Italia, in poche parole, perché ovunque nel mondo l'Italia rappresenta cultura, sviluppo ed eccellenza e permette al nostro Paese di scoprire nuovi orizzonti. La cooperazione culturale contrasta gli stereotipi e i pregiudizi mediante il dialogo e l'apertura mentale. La cultura può e deve essere uno strumento per produrre importanti benefici sociali ed economici all'interno e all'esterno di un Paese. La cultura è un volano di crescita economica non solo nelle sue forme tradizionali, ma anche grazie al crescente numero di aziende che promuovono iniziative culturali, l'innovazione tecnologica e il turismo, attività tipiche delle piccole e medie imprese. Ecco perché le risorse per la promozione culturale rappresentano non una spesa, ma un investimento che favorisce tutti i settori economici di un Paese. Quindi, poniamo la cultura al centro delle relazioni internazionali del nostro Paese e fino a quando questa rimarrà la strada che l'Italia segue, noi del Partito Democratico saremo sempre favorevoli. mi avvio a concludere augurandomi che insieme all'attuazione di questo Accordo vengano promosse iniziative di interscambio economico, anche sotto forma di partenariato e progetti comuni, utili allo sviluppo socio-economico del Laos e all'apertura di nuove opportunità di mercato per l'Italia. Dichiaro, infine, il voto convintamente favorevole del Gruppo Partito Democratico.

è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Repubblica popolare democratica del Laos, soprattutto in ambito culturale, scientifico e tecnologico, incoraggiando anche la collaborazione universitaria, con l'obiettivo di stringere i rapporti bilaterali e di offrire, al contempo, una risposta alla crescente richiesta del Paese asiatico in questi settori. settori prioritari oggetto dell'Accordo sono la scienza di base, l'agricoltura, la tecnologia dell'informazione, la biomedicina, le biotecnologie, l'energia e la conservazione dei beni culturali. Esso rappresenta per l'Italia l'opportunità di allargare i propri orizzonti economici e culturali in Asia. In particolare, l'Accordo afferma la volontà delle due parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti e ricercatori e l'organizzazione di eventi ed esposizioni. La ratifica favorirà certamente gli scambi di esperienze e gli aggiornamenti nel campo delle pubblicazioni e delle traduzioni scientifiche e letterarie. Consideriamo dunque importante, per la crescita del nostro Paese nel Sud-Est asiatico, che si dia attuazione a questo Accordo, volto allo sviluppo economico e culturale e utile alla promozione delle piccole e medie imprese italiane. Il Laos dal 1997 ha optato per l'adesione all'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, avviandosi sulla strada della piena integrazione internazionale; dal 2013 è entrato ufficialmente a far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. La sua economia prevalentemente rurale, che vanta una grande disponibilità di risorse idriche, potrebbe favorire la cooperazione agricola con l'Italia e offrire ulteriori sbocchi economici alle imprese del settore. Anche i comparti idroelettrico e minerario, se si considerano le materie prime di cui è ricco il Paese (in particolare oro, stagno, rame, calcare e gesso), potrebbero far nascere proficue collaborazioni con le nostre imprese. Mi fa piacere che quest'Assemblea, in tema di politica internazionale, abbia dato dimostrazione di piena coesione, nell'interesse ovviamente unico della nostra Italia. Per questi motivi, come già evidenziato anche in Commissione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

e la Repubblica popolare democratica del Laos entrarono a pieno titolo nell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, un'associazione caratterizzata da elevata eterogeneità politica dei Paesi aderenti, ma tuttavia unita da una visione comune dei mercati, nonostante il Laos continui ad avere una forma di governo orbitante su di un partito unico, che richiama, non solo nel nome, il comunismo. Ma del resto l'Oriente e l'Estremo Oriente ormai ci hanno abituati a forme governative inedite. Non è azzardato definire, anche se in scala infinitesimale minore, l'assetto politico-istituzionale di Vientiane simile a quello L'apertura ai mercati è innegabile che abbia portato a risultati di crescita notevoli. Tra il 1985 e il 2017 il PIL è cresciuto di dieci volte, ovvero da un miliardo e 700 milioni di dollari fino a 17 miliardi. Tradotto in termini di reddito *pro capite*, si è passati da 432 a 1.730 dollari. Le stime dell'Economist Intelligence Unit prevedono anche per i prossimi anni margini importanti di crescita. Il *trend* importante, però, non deve oscurare la doverosa e mancata transizione verso un governo plurale. Se da un lato l'attuale sistema comporta un'elevata stabilità e quindi crescita, dall'altro produce un preoccupante grado di corruzione. Non per niente Trasparency international classifica il Laos al 135° posto nel mondo come indice di corruzione percepita. Bisogna però riconoscere che la *leadership* laotiana, nell'ultimo congresso del partito tenutosi nel gennaio del 2016, ha eletto la lotta alla corruzione un'assoluta priorità. Il rafforzamento culturale, politico ed economico con l'Italia, attraverso la ratifica dell'Accordo che oggi trattiamo, ritengo possa agevolare quella trasformazione democratica che tutti auspichiamo. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle esprime il voto favorevole alla ratifica ed esecuzione del disegno di legge n. relativa all'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, sottoscritto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

La giornata di domani sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea, pertanto, tornerà a riunirsi domani alle 18,30 con all'ordine del giorno «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Presidente, nei giorni scorsi Parma, la mia città di provenienza, è stata oggetto di atti che penso meritino la giusta attenzione da parte delle istituzioni e di quest'Assemblea. I muri di uno degli edifici che ospitano l'università, plance pubblicitarie e facciate di edifici privati sono stati malamente imbrattati da scritte con insulti rivolti alle Forze dell'ordine, definite spregevolmente sbirri, e nei confronti di Salvini e Di Maio, i nostri Vice *Premier*, e del senatore Pillon, dichiarando nei loro confronti sentimenti di odio. Da Parma spostiamoci a Roma dove in questa stessa Aula, alcuni giorni fa, un senatore dell'opposizione è intervenuto definendo come atti lesivi della libertà di manifestare e di opinione i necessari controlli da parte delle Forze dell'ordine attuati nei confronti dei manifestanti giunti a Roma sabato 10 novembre e nei confronti di una donna che, sorpresa ad insultare pubblicamente il vice *premier* Salvini, è stata condotta in questura per essersi rifiutata di esibire i documenti a lei richiesti. Controlli che per una certa parte dell'opposizione sono stati infine spunto per un'interrogazione al Ministero dell'interno, sollecitato a far chiarezza su quelle che definirei definirei semplicemente azioni di prevenzione delle Forze dell'ordine per garantire sicurezza nello svolgimento della manifestazione. A fronte di quanto riportato, mi pare che la tanto invocata libertà di pensiero e di manifestare sia intesa a senso unico e che chi non si adegua a un pensiero buonista, permissivo e lassista sia automaticamente bollato in modo negativo e definito fascista, xenofobo, razzista e fomentatore di odio. Mi sento per questo di condannare le incresciose scritte sui muri di Parma, frutto di un indirizzo di pensiero che porta a vedere chi vuole riportare un po' di ordine e dignità in questo nostro Paese in modo negativo e, dall'altra invece, come vittima chi in realtà sta fomentando odio contro le istituzioni e le Forze dell'ordine. Il fatto che la manifestazione sopracitata sia stata definita dalla stessa parte politica intervenuta in quest'Assemblea antirazzista e contro le nuove norme sull'immigrazione la dice lunga. Sinceramente da parte di chi in quest'Assemblea ha invocato la libertà di manifestare e di pensiero in nome della nostra democrazia, vorrei sentire parole di ferma condanna nei confronti di questi gesti che si stanno sempre più ripetendo, non solo a Parma, ma in molte altre nostre città; come a Monza, dove abbiamo letto che «uccidere Salvini non è un reatto», con due «t». Purtroppo è scoraggiante constatare che chi porta avanti il pensiero buonista, permissivo e lassista tende a difendere solo i propri diritti, invocando la Costituzione e condannando proprio chi questa Costituzione l'ha difesa, la sta difendendo e le sta ridando il giusto onore. *(Applausi

di Tempa Rossa, un gigantesco giacimento petrolifero che è stato realizzato in Basilicata, in particolare a Corleto Perticara in provincia di Potenza. Il «Sole 24 Ore» ne parla così: «Là sotto, nel c'è l'iradiddìo di petrolio e di metano». Io aggiungo che c'è anche una montagna decapitata, una torcia alta 130 metri, 840 milioni di barili stimati al ribasso, 15.000 barili al giorno da un solo pozzo di petrolio che è già pronto per essere avviato e altri 60.000 barili al giorno da parte di tutti gli altri pozzi di petrolio. A questo aggiungo ancora i rischi per la salute e per l'ambiente. Questo è Tempa Rossa. Nonostante ciò, il 31 ottobre del 2010, del 2010, 200 maestranze, quasi tutti lucani, hanno perso il posto di lavoro e al 31 dicembre del 2018 altre 600 persone circa perderanno il posto di lavoro, perché Total, o chi per lei, ha detto che non è necessario che chi realizza la pizzeria faccia anche il pizzaiolo. Quindi, queste persone, ragazzi che hanno cullato il sogno di rimanere in Basilicata, padri di famiglia che hanno cullato il sogno di dare un futuro ai propri figli, si vedranno costretti, se Total non cambia registro, a perdere un posto di lavoro, nonostante Total abbia assunto l'impegno formale di formare queste maestranze e quindi avviarle non solo alla costruzione del giacimento petrolifero, ma anche alla sua gestione. Con questo voglio Con questo voglio dire, concludendo, signor Presidente e colleghi, che questo è una battaglia sociale che bisogna combattere con i lavoratori, tra i lavoratori, ma non nell'indifferenza delle istituzioni, per un semplice principio:

colleghi della Lega, ai quali il messaggio è rivolto. Io ho avuto modo in questi giorni, come tutti noi, di essere partecipe al processo che si è svolto qui in Aula,

che non passi, invece, il modello di un partito leghista razzista, che non credo sia nel loro DNA e neanche nelle loro intenzioni. Quindi, richiamo tutti, *in primis* a un comportamento che sia consono e di esempio, perché noi siamo tutti, come sapete, di evidenza pubblica. I

ad essere rispettosi delle regole. Soprattutto, vi ricordo che, prima dei diritti, bisogna avere dei doveri nei confronti di questi ragazzi, trasferendo loro dei modelli di comportamento che siano d'esempio anche per tutti noi.

Leggo una breve riflessione, che ho scritto con Maria Fiore Adami, Presidente della Commissione servizi sociali di Verona, e che così recita: «Chiedere perdono è restituire il posto all'altro. Dargli il diritto di esistere». La frase di Katherine Pancol vuole essere un invito al comico e mentore politico Grillo a chiedere scusa a tutte le famiglie e alle comunità che si impegnano per creare una società in cui i ragazzi affetti dalla patologia dello spettro autistico si sentano accettati e accuditi. A chi si presenta come il *deus ex machina* di una nuova politica basata sulla trasparenza, la legalità e frutto di una democrazia diretta, dico e ricordo che queste poggiano sul rispetto. Il rispetto deve partire dalle parole e spesso le parole feriscono in maniera indelebile. Con il suo siparietto, Grillo ha offeso migliaia di ragazzi e le loro famiglie, con la volontà di sollecitare una risata. Si è dimenticato che ad ascoltarlo c'era una comunità di persone che convive ogni giorno con lo sforzo di togliere lo stigma a questi ragazzi e con l'impegno di integrarli in un mondo che li taccia come diversi; un mondo che, grazie a persone come lei, caro Grillo, alza dei muri e li emargina. Le chiedo di avere rispetto per le persone che vivono con questa patologia disorientati, sperduti in un mondo alternativo a cui si deve offrire sostegno, cura e accoglienza. La vita politica è proprio di coloro che amano stare con le altre persone, non sopra, nemmeno accanto o, peggio, altrove, perché bisogna essere altrove con il proprio cuore per avere l'arroganza di scherzare sulla vita delle persone. Mi chiedo, caro Grillo, chi sarà il prossimo a essere stigmatizzato da lei? Lei, che è il teorico della democrazia a tutti i costi, la aspettiamo mentre in silenzio abbraccia un bambino affetto da qualunque patologia: che le strappi quel sorriso amaro e sprezzante che le incornicia il volto mentre fa i suoi comizi e lo trasformi in qualcosa di più umano, magari in una lacrima di commozione. Il rispetto parte dalle parole, signor Grillo, ma siccome lei è un mago delle parole, dimostri con i fatti che in lei c'è un briciolo di vergogna. Nelle parole e in un gesto di scusa si può realizzare la dignità dell'uomo.

Signor Presidente, signori senatori, il piano di riordino della sanità della Regione Campania ha sancito la chiusura del reparto maternità degli ospedali di Polla e di Sapri, piccoli centri in provincia di Salerno. Se tale chiusura dovesse essere confermata, risulterebbe una ulteriore batosta per questi territori che già vivono situazioni di disagio e di isolamento. L'aria della propria terra e il primo vagito che vuole e deve essere liberato ove sono le proprie radici devono costituire quel filo invisibile a cui rimanere indissolubilmente legati per tutta la vita. Tutto ciò suona come un sinistro viatico; vale a dire: preparatevi a lasciare la vostra terra, i vostri cari, i vostri affetti e le vostre radici ancor prima di nascere, perché qui non c'è presente e neppure futuro. Non basta, signor Presidente, signori senatori, lo spopolamento ormai naturale di questi territori, ma aggiungere la negata possibilità di nascere nei luoghi dove si vive, è veramente troppo. Nella provincia di Salerno insistono paesi che sono antiche perle, autentici scrigni di storia, di cultura, di tradizioni millenarie, incastonati in un paesaggio marino e montano allo stesso tempo, che lasciano, in chi ha il piacere di visitarli e di viverli, anche per poco tempo, sensazioni che non si dimenticheranno mai. Noi non ricerchiamo colpe specifiche o colpevoli. Vogliamo che il diritto di nascere in strutture pubbliche debba essere garantito e custodito in egual modo e misura in tutto il territorio nazionale. Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle vuole dimostrare la propria vicinanza e il proprio sostegno alle future mamme e a tutta la popolazione del Vallo di Diano, affinché tale provvedimento venga al più presto revocato.

Signor Presidente, nella serata di venerdì 16 novembre scorso, unitamente al consigliere regionale Casili, al consigliere comunale Valente e a un gruppo di attivisti e simpatizzanti, ero presente all'interno della sede del Meetup 5 Stelle di Lecce, per presentare l'iniziativa apartitica «Alberi per il futuro», quando due uomini incapucciati hanno fatto irruzione gettando uova ripiene di vernice sui muri e volantini No TAP sul pavimento. Considerata la dinamica del gesto, l'intento era verosimilmente solo intimidatorio e finalizzato a produrre esclusivamente danni materiali. Tuttavia, qualcuno si sarebbe potuto seriamente fare del male se gli schizzi di vernice fossero andati a finire negli occhi e non solo sugli abiti. Ciò che Ciò che fa più male non sono tanto i muri da ridipingere o gli indumenti da buttare, ma proprio quegli schizzi, che nascono da molto lontano e che dovrebbero macchiare nel profondo gli animi e le coscienze di alcuni piuttosto che di altri, quando si dice che l'apparire prevale sull'essere, dimenticando che il silenzio è sovente un atto di responsabilità ed è molto più significativo di molte parole non sufficientemente meditate. La scelta di non enfatizzare determinate vicende in linea con il più elementare buon senso e le linee guida in tema di contrasto agli atti di violenza

nessuna mano si arma da sola e che a scherzare con il fuoco ci si può bruciare. La rabbia è un sentimento prezioso, ma la violenza non genera ragione: essa genera solo altra violenza. La ringrazio, senatore Romano, e mi associo alle sue parole di condanna, al di là del merito e del contenuto, di qualunque episodio di chi vuole impedire ad altri, qualunque sia l'opinione, di esprimere liberamente le proprie idee.

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, fra le molte iniziative memorabili, in senso negativo, della gestione Franceschini del Ministero per i beni e le attività culturali, i dipendenti hanno sofferto e tuttora soffrono specialmente quel decreto ministeriale 23 dicembre 2015 che, disciplinandone il comportamento, proibisce loro di criticare le decisioni dei dirigenti, salvo incorrere in gravi sanzioni. Un caso esemplare delle degenerazioni del decreto bavaglio, come è stato soprannominato, si è verificato in questi giorni in Calabria. La Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio è infatti intervenuta, da Roma, il 12 novembre, per annullare in autotutela la disposizione del soprintendente per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone che avrebbe trasferito d'imperio in San Francesco d'Assisi, da quel giorno, il servizio demo-etno-antropologico già allocato nella sede centrale di Piazza Valdesi, a Cosenza. Sarebbero stati confinati in San Francesco anche un funzionario architetto e il personale afferente, «al fine anche» - scrive il dirigente per motivare il provvedimento - «di garantire l'obbligo della riservatezza»: insinuazione gravissima che non necessita di commento. È quasi superfluo sottolineare che l'autonomia e dunque la discrezionalità riconosciute ad un soprintendente, come ogni forma di potere, presuppongono uno spiccato senso di responsabilità, per non passare dalla discrezionalità all'arbitrio. Arbitrariamente, appunto, e con palese intento ritorsivo, il dirigente cosentino ha tentato di allontanare da sé soggetti colpevoli di non avere appoggiato certe sue scelte non per mera divergenza di opinioni, ma perché discutibili sul piano della correttezza amministrativa. Mi riferisco soprattutto alle grandi opere pensate per Cosenza dal sindaco e disinvoltamente condivise dal soprintendente. Alcuni di loro avevano anche svolto, forse colpevolmente agli occhi del dirigente, attività sindacale. L'intervento provvidenziale del direttore generale ha bloccato, come dicevo, il trasferimento coatto e imposto l'annullamento della condanna all'esilio per i dissenzienti. In generale, ritengo sia ora di restituire dignità alla funzione di dirigente MIBAC e ai ruoli subordinati, abrogando quel cosiddetto decreto bavaglio che alcuni, come ho appena dimostrato, usano quale mezzo di rappresaglia per poter consumare vendette personali che nulla hanno a che vedere con i compiti delicatissimi di un soprintendente. Chiederò al ministro Bonisoli di valutare seriamente l'ipotesi appena avanzata e invoco, nel farlo, il concorso di tutti i colleghi. In questa stagione obiettivamente crepuscolare per il MIBAC, gravemente depotenziato dalla pessima riforma del precedente Ministro, il libero pensiero (anche critico) di professionisti con decenni di esperienza non deve esporli a fare la fine «*de l'abbacchio ar forno»*, ma va se mai incoraggiato ad emergere. È un patrimonio al quale non si può e non si deve rinunciare, se si vuole sperare di rivitalizzare quello che altrimenti finirà per assumere, in via definitiva e irreparabile, la sostanza e la forma di una scatola bella ma vuota. *(Applausi dal

colleghe e colleghi, il 18 novembre 2013 il ciclone Cleopatra si è abbattuto sul territorio gallurese in Sardegna, uccidendo diciannove persone, di cui nove nella sola città di Olbia: Morgana (due anni) e la mamma, Enrico (quattro anni) con il papà, Anna e Maria nelle loro case, Bruno, Sebastiana e Maria risucchiati da una voragine creatasi nel manto stradale. Interi quartieri sono stati spazzati via da un'onda altissima di acqua e di fango. Tanta la solidarietà dei cittadini sardi, ma pochi i risarcimenti agli ingenti danni subiti dalle vittime dell'alluvione e al momento nessuna giustizia per le famiglie, con ipotesi di reato già a rischio prescrizione. Pochissimo è stato fatto per mettere in sicurezza il territorio gallurese: è solo di pochi mesi fa l'inizio dei lavori da parte dell'ANAS per eliminare la voragine che ha inghiottito tre persone, un ponte è stato abbattuto e da poco ricostruito più alto. Tuttavia, tante sono le opere ancora necessarie. Intanto la politica discute sul piano di mitigazione del rischio idrogeologico, anzi su due piani: uno è fermo in sede di valutazione di impatto ambientale, l'altro è uno studio di fattibilità che sostiene il contrario del primo. L'amministrazione comunale vorrebbe risolvere il problema dovrebbe trasformare i cittadini in esperti di ingegneria idraulica. Intanto la città, che nel frattempo ha subito anche l'alluvione del 2015, vive nel terrore che il fiume si ingrossi e si ripeta la tragedia del 2013. Faccio un appello al buon senso di tutti gli amministratori locali, della Regione Sardegna e del ministro Costa, affinché si pensi solo ed esclusivamente al bene della comunità gallurese e si intervenga il più presto possibile per attuare un vero e proprio piano antialluvione.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

Grazie a tutti.